la possibilità che un gruppo di sottufficiali e ufficiali dei ROS dei carabinieri si sarebbe recato nel carcere americano di Guantanamo - tra l'altro tristemente famoso per l'intervento di tutte le organizzazioni internazionali - ad interrogare non si sa chi e non si sa per mandato di chi. chi. Il fatto di per sé è gravissimo perché, stando alle notizie raccolte, che derivano da un interrogatorio avvenuto durante un dibattimento processuale di uno di questi ufficiali dei ROS, ovviamente ricevuto alcun mandato e pare che solo *ex post* avrebbero riferito alcune informazioni a sostituti procuratori di Torino, i quali non si capisce quale uso ne abbiano fatto. Ora, ovviamente,

i processi si svolgono sui giornali; processi a senso unico, che non tengono conto del fatto che, ancora oggi, ma ancor più nel 2002, la situazione internazionale era tale da richiedere un'attività investigativa che probabilmente è restata nell'ambito della legalità. Non mi risulta, infatti, che per procedere ad interrogatori occorra di volta in volta chiedere autorizzazioni o

Senatore Martone, per cortesia.

che vi è una parte politica (probabilmente la maggior parte di questo Parlamento) che non la pensa esattamente nello stesso senso. Ben vengano i chiarimenti e gli approfondimenti, ma i processi non si devono svolgere né sulla stampa e nemmeno,

L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine ad disegno di legge n. 772 recante: «Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali», collegato alla manovra di finanza pubblica. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

sentito il rappresentante del Governo -, osserva che il disegno di legge rispetta il termine di presentazione del 15 novembre previsto dalla legislazione vigente e che la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 approvata con risoluzione dall'Assemblea del Senato l'11 ottobre 2006, qualifica espressamente il suddetto provvedimento come "collegato" alla manovra di bilancio 2007. Rileva inoltre che il provvedimento è omogeneo nel suo contenuto e nelle sue finalità complessive ed è inquadrabile, complessivamente e nelle singole parti che lo compongono, nella materia della promozione della concorrenza, indicata dal Documento di programmazione economico-finanziaria nell'ambito delle politiche della crescita di cui al capitolo IV.1, ove sono espressamente richiamati i servizi pubblici locali come uno dei settori prioritari di intervento. Tali indicazioni appaiono quindi coerenti con le finalità del disegno di legge collegato posto che, in base al disposto dell'articolo 1, esso mira "al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni"».

preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente, nonché dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento, così come approvati dalle risoluzioni parlamentari.

l'esame parlamentare del rendiconto generale dello Stato consente la verifica, *a**posteriori*, da parte del Parlamento, nella forma della legge, dell'avvenuto rispetto di quanto autorizzato con la legge di bilancio ai fini di un'ordinata gestione finanziaria È utile altresì rammentare che il rendiconto non può dare conto compiutamente dei flussi annuali di spesa ed entrata e della variazione delle consistenze di attività e passività patrimoniali per tutto il settore delle pubbliche amministrazioni, ove confluiscono enti pubblici diversi dallo Stato centrale. Il rendiconto, come analiticamente esposto in relazione, fotografa la difficile fase congiunturale dell'economia italiana dell'anno 2005, che ha comportato un peggioramento complessivo dei conti dello Stato: un

un andamento delle spese correnti in continuo aumento, che non ha però comportato effetti benefici sulla nostra economia; una politica tributaria caratterizzata da misure *una* *tantum* (ad esempio condoni) che non ha raggiunto i risultati preventivati. Anche in relazione al rendiconto per il 2005 va segnalato come l'attuazione del disegno di programmazione e controllo insito nella legge n. 94 del 1997 sia ancora in fase di attuazione. Sul piano più generale, peraltro, va ricordato che l'applicazione del modello di riforma fondato sul principio della programmazione per obiettivi necessiterebbe dell'introduzione di indicatori di prodotto e di impatto all'interno delle note preliminari di bilancio coerenti con le direttive generali di inizio d'anno. Passando ai risultati differenziali, si rileva come nel 2005 si conferma il divario tra i dati di previsione e i risultati definitivi della gestione di competenza delle entrate e delle spese che, scontato del tasso storicamente fisiologico, appare tuttavia significativo in relazione alle entrate extratributarie, alle spese correnti e alle partite finanziarie. I saldi complessivi mostrano un risparmio pubblico di competenza di gestione positivo di soli 1.509 1.509 milionidi euro, a fronte di un analogo dato pari a 15.217 milioni di euro nel 2004, con un miglioramento, tuttavia, di 28.529 milioni sulle previsioni definitive. Il saldo netto da finanziare si attesta a 35.210 milioni, milioni, in netto peggioramento rispetto ai 21.156 milioni del 2004, ritornando in sostanza sui livelli registrati nel 2003. Il ricorso al mercato finanziario mostra un risultato 2005 che si attesta a 203.523 milioni di euro, in calo marginale rispetto ai 214.084 del 2004, scontando un miglioramento di 56.406 milioni rispetto alle previsioni definitive dell'anno. Si nota che il documento in esame contiene anche un'analisi delle spese finali per funzioni-obiettivo, che evidenzia come i servizi generali delle pubbliche amministrazioni abbiano assorbito il 48,43 per cento (era il 46,46 per cento nel 2004) degli impegni relativi alle spese finali, seguiti dalla protezione sociale, dagli affari economici e dall'istruzione. Utili informazioni - leggendo i documenti - sono altresì ritraibili dai dati ricavati dall'analisi economica delle spese finali,

una continua crescita della spesa corrente mentre quella in conto capitale, per 46.794 milioni di euro (era 47.364 milioni di euro nel 2004) è in calo, anche in tale ambito confermandosi pertanto la dequalificazione della spesa pubblica. Passando ai dati della gestione di cassa del bilancio dello Stato per il 2005, si sottolinea il notevole peggioramento del risparmio pubblico al lordo delle regolazioni contabili, che è passato dai meno 603 milioni di euro del 2004 a un dato negativo di 16.414 milioni. Il saldo netto da finanziare lordo si evidenzia per il 2005 con un valore di 48.836, anch'esso in peggioramento rispetto ai 33.587 milioni di euro del 2004. Il ricorso al mercato si attesta, in valore assoluto, al lordo delle regolazioni contabili, a 222.853 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al dato relativo al 2004 e in miglioramento di circa 74.000 milioni rispetto alle previsioni definitive. Passando ai dati della gestione in conto residui del bilancio dello Stato per il 2005, si può notare come tale conto, in relazione ai valori esposti al 1° gennaio 2005 e quindi in relazione alle risultanze riferibili alla gestione degli esercizi precedenti, presenti un'eccedenza passiva, come saldo tra residui passivi, per 121.294 milioni di euro, ed attivi, per 116.856 milioni di euro, pari a 4.438 milioni (nel 2004 tale eccedenza si mostrava attiva per 23.628 milioni di euro). Nel corso dell'esercizio 2005 la revisione di tali dati ha portato ad accertare residui attivi per 122.959 milioni e passivi per 110.180, con un'eccedenza attiva pari a 12.779. Si segnala quindi una sostanziale difficoltà a tenere sotto controllo i residui attivi e passivi. Al 31 dicembre 2005 il totale complessivo dei residui attivi (tenuto conto quindi anche degli effetti della gestione relativa alla quota residui degli esercizi precedenti) è stato pari a 151.247 milioni di euro, in corrispondenza a 108.662 milioni derivanti dagli anni precedenti e a 42.585 milioni maturati nel 2005, e quello dei passivi a 119.138 milioni di euro, in corrispondenza a 65.879 milioni rimasti dagli anni precedenti e a 53.259 milioni maturati nel 2005. Si sottolinea il dato costituito dalla sempre più rilevante quota di residui attivi proveniente dagli esercizi pregressi, il cui ammontare necessiterebbe di un'accurata valutazione in ordine alla loro effettiva esigibilità. Passando al conto generale del patrimonio dello Stato per il 2005, si fa presente come l'eccedenza passiva si è attestata a 1.354 miliardi, a fronte dei 1.338,8 del 2004 e dei 1.306,7 miliardi del 2003, confermando la tendenza al peggioramento della situazione patrimoniale dello Stato, peggioramento ascrivibile, per il 2005, al consistente peggioramento della passività, ormai prossima al valore dei 2.000 miliardi di euro, solo parzialmente compensato dall'aumento per 67 miliardi di euro delle attività. Nel dettaglio, le attività finanziarie, che rappresentano l'82,4 per cento del totale, si assestano nel 2005 a 494.547 milioni di euro, con un incremento di 61.981 milioni e si attestano nel 2005 a 1.953.594 milioni di euro. Tale ultimo dato è connesso anche ad un notevole incremento nei debiti di tesoreria, passati da 561.000 milioni circa di euro a 617.000 milioni per cui la situazione del Tesoro risulta, nel complesso, peggiorata, con un saldo di meno 27.612 milioni di euro. In sede di Commissione è stata osservata la necessità di analizzare in maniera più compiuta le cause degli scostamenti tra previsioni e dati effettivi di spesa, al fine di ridurre il più possibile il fenomeno negativo e patologico delle eccedenze

dei singoli Ministeri, dove è specificato che le eccedenze, determinatesi in 740 milioni di euro nel conto di competenza, in 3 milioni in quello dei residui e in 799 milioni in termini di cassa, derivano sostanzialmente da spese i cui pagamenti vengono eseguiti con modalità del tutto particolari, quali quelle per la gestione di spesa attraverso l'emissione di ruoli di spesa fissa e che per le spese gestite con ruoli di spesa fissa i pagamenti vengono invece contabilizzati solamente dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, generando talvolta un esubero in occorrenza rispetto alla previsione, con il conseguente formarsi della eccedenza. È opportuno evidenziare, poi, il dato negativo dell'inversione del percorso registrato negli ultimi anni, in cui era emersa una sensibile riduzione del finanziamento della gestione di bilancio da parte della gestione di tesoreria, che denota una rinnovata criticità nella coordinazione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione delle delle previsioni iscritte in bilancio. Va ricordato, in relazione al rendiconto dell'entrata, che la Corte dei conti ha segnalato - bisogna, secondo me, segnalarlo anche in questa sede - una serie di elementi incongrui, sia contabili che interni al rendiconto, nonché dedicato un'apposita appendice alle problematiche inerenti l'attendibilità e l'affidabilità dei dati contabili (un elemento, quindi, preoccupante che sottopongo all'attenzione del Parlamento), in merito alle quali si segnalano gli effetti contabili correlati all'abrogazione dell'obbligo di versamento da parte delle banche, entro fine anno, dell'1,5 per cento delle somme riscosse nel 2003. 2003. La Corte dei conti ha altresì evidenziato come sia necessario avere informazioni più esaustive in relazione al fenomeno delle regolazioni contabili e debitore, sia in termini di raccordo con i pertinenti capitoli che ai fini di un'illustrazione delle cause alla base della loro formazione. Pur riconoscendo che l'esame del disegno di legge di rendiconto non rappresenta il momento più adatto per una valutazione dei saldi di finanza pubblica riferiti al complesso delle pubbliche amministrazioni, occorre sottolineare l'utilità di una sintetica valutazione sul punto. Si evidenzia, innanzitutto, l'ulteriore peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (elemento che, ricordo, è rilevante ai fini dei parametri europei), passato dal 3,4 per e 2004 al 4,1 del 2005, principalmente per effetto dell'aumento della spesa corrente alla quale è altresì ascrivibile, stante la sostanziale stabilità delle entrate fiscali, l'ulteriore decremento dell'avanzo primario, ormai quasi azzeratosi rispetto al livello della precedente legislatura, quando si era attestato su livelli tali da garantire la sostenibilità del processo di rientro del debito pubblico, che, infatti, è aumentato in rapporto al PIL, passando dal 103,9 cento del 2004 al 106,4 nel 2005. In termini più generali, si segnala, infine, sempre in relazione al comparto delle pubbliche amministrazioni, il peggioramento della posizione debitoria degli enti territoriali e la scarsa efficacia dei provvedimenti di contenimento della spesa concepiti in termini di tetti o tagli percentuali uniformi, operati in assenza di interventi sulla legislazione sostanziale. Qui, com'è noto, interviene la finanziaria del 2007, operando un cambiamento, perché si interviene sui saldi, così com'è noto che,

gentili colleghi e gentili rappresentanti del Governo, in relazione al disegno di legge di assestamento in esame si segnala, per quanto di competenza, che tale strumento giuridico-contabile ha mantenuto inalterata la propria configurazione tecnico-giuridica, nonostante il dibattito sulla sua insufficienza rispetto alle esigenze di controllo e correzione degli andamenti di finanza pubblica. Allo stato attuale, esso rimane uno strumento per l'aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge; si connette funzionalmente con il disegno di legge del rendiconto relativo all'esercizio trascorso, dal quale si evince l'entità effettiva dei residui alla data del 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti di bilancio vengono adeguati in relazione alle previsioni di gettito, collegate alle grandezze economiche ed alla attività di accertamento. Per quanto riguarda le spese, quelle aventi carattere discrezionale sono adeguate a nuove e diverse esigenze intervenute, mentre per la determinazione delle autorizzazioni di pagamento gli stanziamenti vengono adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Entrando nel merito del provvedimento, si osserva che le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2006 presentavano inizialmente un peggioramento dei saldi di bilancio al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio. L'approvazione di un emendamento del Governo in prima lettura alla Camera ha poi invertito il segno dell'impatto dell'assestamento sui saldi di bilancio di competenza, determinandosi pertanto un miglioramento degli stessi. In particolare, il disegno di legge iniziale recava un peggioramento di 1.800 milioni di euro del saldo netto da finanziare, che raggiungeva i 38.464 milioni di euro. La quota di incremento ascrivibile alle variazioni per atto amministrativo è quasi interamente riconducibile alla riassegnazione alla spesa di maggiori somme affluite in entrata nel 2005, mentre quella relativa alle proposte di assestamento, pari a 1.487 milioni di euro, deriva quasi interamente dalle maggiori spese correnti. Anche l'avanzo primario e il risparmio pubblico presentavano un peggioramento, rispettivamente di 1.506 e 1.482 milioni di euro, inclusi gli effetti degli atti amministrativi. Il ricorso al mercato presentava un incremento di 2.929 milioni, quasi interamente ascrivibile alle proposte di assestamento, collocandosi sul livello complessivo di 259.559 milioni di euro. Da un punto di vista metodologico, si sottolinea come il peggioramento dei saldi appena evidenziato offra l'opportunità per una riflessione in rapporto alla funzione propria del disegno di legge di assestamento, ovvero se, a fronte degli indicati aumenti, anche se in dipendenza di spesa in parte obbligatoria, non si debba fare il possibile in vista della riduzione della quota discrezionale della spesa. Si segnala anche il fatto che sull'andamento della spesa ha inciso, peraltro in maniera significativa, anche il decreto-legge n. 194 del 2002 (cosiddetto decreto taglia spese), convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002. Per tali spese, riguardanti generalmente benefici assimilabili a diritti soggettivi - peraltro già utilizzati dai beneficiari - ovvero spese aventi natura obbligatoria, si è verificata la necessità di rifinanziarle con appositi provvedimenti legislativi di carattere sostanziale in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2007. Si osserva al riguardo che questa decisione, peraltro attuativa del citato decreto-legge taglia spese, ripropone una serie di problemi già evidenziati negli anni passati (anche in sede di assestamento), in particolare in relazione alla trasformazione - avvenuta ad opera dello stesso decreto taglia spese - in tetti di spesa degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato sulla base della legislazione vigente, allorquando questa reca previsioni di spesa corrispondenti ai cosiddetti oneri inderogabili. Merita inoltre di essere sollevata la questione, connessa all'indicato aumento delle spese correnti, del grado di efficacia delle misure di contenimento della spesa recate dalla legge finanziaria per il 2006, ivi compreso il funzionamento della regola del tetto di crescita per alcune categorie di spesa, fissato nel 2 per cento Per quanto concerne le variazioni proposte con il provvedimento di assestamento, si rileva che il citato incremento delle spese correnti è ascrivibile ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per circa 1.750 milioni (di cui circa 900 a favore dei Comuni e circa 800 a favore delle Regioni), ai consumi intermedi per 670 milioni e ai redditi da lavoro dipendente per 490 milioni. Le spese in conto capitale denotano una riduzione, sia a livello di contributi alle amministrazioni pubbliche, per 136 milioni, che per gli investimenti fissi lordi, per 32 milioni; aumentano invece i contributi alle imprese, per 225 milioni. Al riguardo il Governo in Commissione ha chiarito che gli incrementi di spese correnti disposti con il provvedimento in esame sono dovuti a oneri di carattere obbligatorio, mentre l'efficacia della manovra 2006 potrà essere verificata solo a consuntivo. Per quanto concerne le entrate, in aumento, tale dato deriva per 2.000 milioni dalla revisione delle stime operata dalla *due* *diligence* per il comparto tributario e per 132 milioni da altre entrate; dall'analisi dello stato di previsione dell'entrata si evince che la maggior parte dell'aumento complessivo delle entrate tributarie risulta ascrivibile alle imposte sostitutive (per 900 milioni). Gli altri aumenti derivano dall'IVA su scambi interni e intracomunitari (per 300 milioni) e dall'IVA su importazioni (per 200 milioni). Aumentano poi anche le previsioni di entrata per altri introiti diretti (300 milioni) e indiretti (200 milioni). Questi ultimi si riferiscono all'imposta di bollo. In relazione alla composizione e alle determinanti delle maggiori entrate inserite nell'assestamento in seguito alla *due* *diligence*, ci si sofferma in particolare sugli altri introiti diretti. Si tratta dell'unità previsionale di base 1.1.7.2, che si riferisce alle entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul reddito. Si segnala sul punto che il Governo in Commissione ha chiarito che la revisione delle stime di entrata del capitolo 1200, inserito nella suddetta unità previsionale di base, è correlata a una valutazione complessiva del recente andamento del gettito che affluisce su tali capitoli, prescindendo da un'analisi puntuale delle singole componenti del gettito predetto che, a motivo della varietà e residualità delle stesse, si presenterebbe difficoltosa e non sufficientemente attendibile. Interamente ascrivibili, poi, alle proposte di assestamento dal lato della spesa corrente sono le variazioni relative alle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, pari a 1.264 milioni di euro, mentre non sono registrate operazioni - sempre ovviamente a titolo di regolazioni debitorie - relativamente alle entrate. Si osserva quindi che, anche in termini di cassa, il disegno di legge di assestamento determina un peggioramento, al netto delle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, del saldo netto da finanziare, che aumenta infatti da 65.538 milioni a 67.598 milioni, con un differenziale pari a 2.060 milioni, corrispondente al 3,14 per cento. In corrispondenza con il saldo netto da finanziare peggiora anche l'avanzo primario, nella misura di 1.719 milioni (di cui 754 milioni per atti amministrativi), quindi del 29 per cento circa. Il risparmio pubblico, di segno negativo, migliora invece di 1.027 milioni (tenuto conto di un effetto positivo di 2.670 milioni per atti amministrativi), con un peggioramento dovuto all'assestamento di 1.643 milioni: l'effetto netto è quello di un miglioramento del 3,25 per cento. Il ricorso al mercato, infine, si incrementa per 4.636 milioni (di cui 2.224 milioni per atti amministrativi), aumentando dell'1,77 per cento. Al riguardo, rilevato che le variazioni per atto amministrativo impattano negativamente sul saldo netto da finanziare e positivamente sul risparmio pubblico, sarebbe utile acquisire il dettaglio delle operazioni alla base di questa divergenza, atteso che la relazione illustrativa richiama in merito unicamente i trasporti di titoli di pagamento insoluti (per 1.911 milioni). Anche per la cassa, poi, sono interamente ascrivibili alle proposte di assestamento dal lato della spesa le variazioni relative alle regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA, che aumentano di 1.264 milioni di euro, attestandosi sui 59.795 milioni di euro complessivi. Analogamente, non si registrano operazioni - sempre ovviamente a titolo di regolazioni debitorie - relativamente alle entrate. Si ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati il Governo ha depositato una tabella recante la sintesi degli effetti delle proprie proposte emendative, specificando che, rispetto ai saldi del disegno di legge di assestamento, si è tenuto conto di una ulteriore regolazione debitoria in conto capitale, riguardante i disavanzi delle ASL e pari a 1.383 milioni. Al riguardo, sarebbe opportuna una delucidazione in merito alle motivazioni che hanno determinato il cambiamento di classificazione della posta, nonché la specifica natura della stessa. Sul punto si rileva che tale modifica potrebbe essere connessa al fenomeno dell'accumulo di debiti da parte delle ASL, che vengono in gran parte ripianati *ex post* dallo Stato centrale, per quanto ciò si verifichi prevalentemente con riferimento alle spese correnti, mentre quella in parola è spesa in conto capitale. A tale proposito il Governo in Commissione ha chiarito che la regolazione debitoria in questione è classificata come «Altri trasferimenti in conto capitale alle Regioni». Passando poi ai residui, si precisa che i residui passivi accertati al 31 dicembre 2005, al netto di quelli relativi al rimborso prestiti (pari a 3.334 milioni), ammontano a 115.804 milioni, dei quali 49.990 milioni derivano dalla gestione 2005. L'importo dei residui di nuova formazione, pari, al netto del rimborso prestiti, a 49.990 milioni, è composto per 29.578 milioni da residui di parte corrente, mentre 20.412 milioni sono relativi alle spese in conto capitale. Per la spesa corrente, essi riguardano in prevalenza i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (17.174 milioni di cui 7.517 alle Regioni). Per quanto concerne i nuovi residui in conto capitale, essi sono costituiti in gran parte dai contributi alle imprese (oltre 4.500 milioni) e da altri trasferimenti in conto capitale (4.422 milioni). Lo scostamento per singolo Ministero verificatosi fra i residui passivi presunti al 1° gennaio 2006 e quelli accertati in sede di rendiconto 2005 è collegato soprattutto ai maggiori residui accertati in relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze (52.572 milioni), del lavoro (2.316 milioni) delle infrastrutture e trasporti (3.168 milioni). Lo scostamento dei residui accertati rispetto ai residui presunti risulta essere il più ingente dal 1996, raggiungendo il valore del 117 per Sulle cause di un tale andamento sarebbe utile avere qualche ulteriore delucidazione dal Governo. Infatti, solo nel 2003 i residui accertati hanno superato il valore di quelli presunti per una percentuale molto elevata, decisamente superiore rispetto a quella degli anni precedenti e comunque comparabile solamente con gli scostamenti registrati prima del 1997. Quest'anno il disegno di legge fornisce altresì nuove informazioni sui residui passivi, classificandoli in 3 categorie anche in funzione dell'impatto (diretto, indiretto o nullo) che si può determinare sul conto economico delle In particolare, i residui connessi a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche e a fondi da ripartire determinano un effetto sui saldi più diluito nel tempo, in quanto l'effetto stesso viene registrato sul conto della pubblica amministrazione nel momento dell'effettivo prelievo dalla tesoreria. Una serie storica riportata nel disegno di legge di assestamento - riferita agli anni dal 1995 al 2005 - mette in evidenza un andamento sostanzialmente costante dei residui con impatto diretto sulla pubblica amministrazione, che denota quindi l'esistenza di fattori strutturali alla base della formazione degli stessi; ugualmente, i residui non aventi impatto presentano un andamento relativamente costante nel tempo. Per quanto riguarda invece i residui con effetto indiretto sull'indebitamento netto, si verifica una crescita in valore assoluto dai 18 miliardi circa del 1995 ai 76 miliardi circa degli esercizi dal 2000 al 2002; negli esercizi dal 2003 al 2005, invece, il livello scende al di sotto dei 60 miliardi. Tale andamento viene ricondotto alle misure finalizzate al controllo di cassa attuate dal Tesoro a partire dal 1996, in quanto l'incremento dei residui passivi è stato determinato anche dalla riduzione delle disponibilità di tesoreria dei diversi enti. Conseguentemente, sono aumentati i residui passivi sul bilancio dello Stato, ma si sono ridotti i debiti della tesoreria nei confronti degli altri soggetti pubblici. L'analisi dell'incidenza sul prodotto interno lordo delle tre categorie di residui sopra individuate denota quindi un andamento relativamente stazionario nella serie storica relativa ai residui con effetti diretti e nulli sul conto della pubblica amministrazione, mentre quelli con effetti indiretti mostrano una dinamica accentuata nel periodo (1996-1998) corrispondente a forti strette di cassa, per discendere poi progressivamente dal 2001 in avanti. A questo proposito, si ricordano alcune importanti modifiche intervenute dal 1997 ad oggi con riferimento alle modalità di accreditamento dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali; si tratta, in particolare, del cosiddetto sistema di monitoraggio, che prevede che i pagamenti a carico dello Stato a favore di Province e Comuni vengano effettuati al raggiungimento di limiti di giacenza predeterminati e dei limiti ai prelevamenti dai conti e dalle contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, nella misura del 2 per cento in più rispetto ai prelevamenti dell'anno precedente; i destinatari sono quasi tutti soggetti titolari di conti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria statale, inseriti nell'elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2005, ad eccezione degli enti interessati dal Patto di stabilità interno. Al riguardo, il Governo in Commissione ha chiarito che presumibilmente gli effetti dei residui sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione per il 2006 saranno in linea con quelli registrati nel 2005, pur in presenza di una massa di residui più elevata. Con riferimento all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, nel disegno di legge di assestamento viene fissato il limite di 66.500 milioni di euro, con un aumento di 6.500 milioni di euro rispetto all'importo determinato nella legge di bilancio che lo indicava in 60.000 milioni. Al riguardo, in Commissione il Governo ha chiarito che detto aumento del limite massimo di emissione dei titoli pubblici era correlato a precedenti stime di revisione al rialzo del fabbisogno di cassa del settore statale. Solo successivamente sono intervenuti più positivi andamenti del fabbisogno, che hanno dato luogo alla revisione effettuata da ultimo nella Nota di aggiornamento del DPEF 2007-2011 e nella Relazione previsionale e programmatica per il 2007. Come anticipato, si rappresenta che la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, ha approvato un emendamento del Governo, le cui variazioni riguardano unità previsionali di base sia di entrata che di spesa. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare (in termini di competenza) scende a 35.544 milioni, con un miglioramento di circa 3.920 milioni rispetto al disegno di legge iniziale; il risparmio pubblico migliora di 4.761 milioni, passando ad un valore negativo di 3.098 milioni; il ricorso al mercato passa a 231.675 milioni, con una diminuzione di 3.920 milioni. L'emendamento determina quindi, per i citati saldi, un miglioramento anche con riferimento alle previsioni contenute nella legge di bilancio. In termini di cassa, l'effetto positivo di oltre 1.500 milioni recato dall'emendamento predetto determina un miglioramento rispetto alla legge di bilancio con riferimento al saldo netto da finanziare ed un contenimento del peggioramento in relazione al ricorso al mercato. Peraltro, era stata già anticipata la possibilità dell'introduzione di apposito emendamento, in quanto non tutti gli elementi necessari per una quantificazione puntuale del gettito dell'esercizio finanziario 2006 erano disponibili; in particolare, con riguardo al comparto tributario, non erano ancora noti i dati concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, il che pone il problema più generale della congruità del termine di presentazione del disegno di legge di assestamento al 30 giugno. Tale emendamento al disegno di legge ha inoltre lo scopo di allineare le previsioni di bilancio assestate con il contenuto del DPEF per gli anni 2007-2011, mentre non tiene conto delle modificazioni da apportare in conseguenza del riordino dei Ministeri, né degli effetti derivanti dal decreto-legge n. 223 del 2006, che formeranno oggetto di appositi decreti di variazione al bilancio. Al riguardo si ricorda che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del decreto-legge n. 181 del 2006, riguardante il riordino dei Ministeri, il Governo aveva accolto un ordine del giorno contenente l'impegno a procedere in un'unica sede, possibilmente in occasione dell'esame del disegno di legge di assestamento, all'adeguamento dell'articolazione del bilancio dello Stato in relazione al riassetto delle amministrazioni, mentre sembra prefigurarsi un'attuazione del suddetto impegno demandata ad atti di natura meramente amministrativa, destinati a riflettersi evidentemente sulla struttura del bilancio a partire dal 2007. Un'altra questione sollevata in Commissione riguarda il mancato recepimento degli effetti della sentenza europea in materia di IVA. Nella Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 il Governo ha quantificato l'impatto negativo sul gettito in 3,7 miliardi per il 2006 e, in ragione della competenza economica, in 13,4 miliardi per la corresponsione degli arretrati. Al riguardo il Governo durante l'esame in Commissione ha chiarito che non si prevedono corrispondenti variazioni ai fini del saldo netto da finanziare di competenza e di cassa relativo all'anno 2006. Ciò in considerazione dei diversi criteri di contabilizzazione di tali poste ai fini del disegno di legge in esame, in cui le previsioni sono costruite in termini di contabilità finanziaria competenza giuridica e cassa - e non di competenza economica, come invece quelle contenute nel DPEF e nella relativa Nota di aggiornamento. Tornando all'illustrazione dell'emendamento, per quanto riguarda le unità previsionali di entrata le variazioni positive più ingenti si riscontrano nelle entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione dell'IRE per circa 3.618 milioni, dell'IRES per circa 2.495 milioni, delle imposte sostitutive per circa 2.493 milioni, dell'IVA su scambi interni ed intracomunitari per circa 2.080 milioni e dell'IVA sulle importazioni per 1.148 milioni. Variazioni negative significative si rilevano invece con riferimento alle entrate derivanti da Lotto e lotterie (meno 1.349 milioni alle imposte sui generi di monopolio (meno 633 milioni) e agli altri introiti diretti (meno 531 milioni). Si riscontrano due ulteriori variazioni di segno negativo che riguardano le entrate extra-tributarie: si tratta di quelle derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti per minori 500 milioni e di quelle relative ai prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari per 2.500 milioni. Questi ultimi, in particolare, si compongono di 1.500 milioni riferiti al capitolo 2368 (Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze) e 1.000 milioni riferiti al capitolo 3342 (Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria), di cui 500 milioni con riferimento all'articolo 1 (Versamento da parte dell'INPS dei contributi di malattia riscossi) e 500 milioni con riferimento all'articolo 15 (Altri introiti eventuali). Con riferimento alla ingente variazione negativa inerente al capitolo 2368, il Governo, in Commissione, ha chiarito che è stata apportata al fine di adeguare la previsione all'andamento del gettito del capitolo in esame, che porta a prevedere entrate per l'anno 2006 inferiori a quelle previste con la legge di bilancio, data la natura promiscua di tale voce di bilancio. Si ricorda che il rappresentante del Governo ha affermato che talune maggiori entrate hanno carattere senz'altro non strutturale, quali ad es. le imposte sostitutive sulla rivalutazione degli immobili delle imprese. Carattere non strutturale rivestono inoltre le maggiori ritenute le maggiori ritenute IRPEF legate alla circostanza che alcuni aumenti derivanti da rinnovi contrattuali sono stati erogati nel corso dell'anno. In relazione ad altre entrate, quali quelle legate al rapporto fra l'imposizione sul reddito delle persone fisiche e il *fiscal* *drag*, nonché l'imposizione ai fini dell'IVA, il rappresentante del Governo ha affermato l'impossibilità, per il momento, di valutare se tali effetti siano o meno strutturali. Al riguardo, si sottolinea che appare opportuno acquisire chiarimenti più specifici su quanta parte del maggiore gettito accertato abbia natura strutturale e quanta parte sia dovuta principalmente all'attuale fase di espansione ciclica dell'economia. Ciò per valutare in che misura tali maggiori entrate possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale della pubblica amministrazione (cioè quello corretto per gli effetti del ciclo), valutazione resa necessaria dalla circostanza che gli impegni di rientro dal *deficit* assunti dal nostro Paese in sede europea riguardano l'aggiustamento del saldo di bilancio al netto del ciclo e delle *una* *tantum*. Su questo punto le nuove previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF 2007-2011 danno conto di circa 6 miliardi di maggiori entrate per il 2006, di cui circa 5 miliardi sono stati considerati strutturali e proiettati al 2007. In quella sede le entrate vengono peraltro contabilizzate sulla base del criterio della competenza economica. Con riferimento alla spesa, il rappresentante del Governo ha specificato che si intende provvedere, in relazione al finanziamento della missione italiana in Libano, ad una variazione di bilancio che registrerà un incremento delle entrate pari a 400 milioni, a fronte di un incremento di 220 milioni, con un beneficio sui saldi di bilancio di circa 180 milioni. Analoga circostanza è stata infatti confermata in sede di Commissione bilancio presso il Senato. Al riguardo, si ricorda che le maggiori entrate in questione sono state utilizzate per la copertura finanziaria del decreto-legge n. 253 del 2006 (Atto Senato n. 1026), relativo appunto alla missione in Libano, sulla base dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 266 del 2005 Tale norma regola l'utilizzo delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio per la copertura finanziaria di oneri associati a situazioni di carattere straordinario indicate nella norma stessa. Conclusivamente, nel prendere atto della positiva novità delle maggiori entrate tributarie accertate, si rileva comunque come non si possa prescindere dall'affrontare con estremo rigore la manovra di finanza pubblica per il 2007, in modo da operare gli interventi necessari al recupero della competitività del Paese. L'importo delle maggiori entrate accertate rende infatti la situazione dei conti pubblici meno pesante, ma non fa venir meno le ragioni di un rigoroso e coerente comportamento da tenere a salvaguardia della finanza pubblica, per la crescita del Paese e per l'equità sociale, ove si consideri lo scostamento registrato in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario 2005, tra le previsioni definitive ed i risultati di gestione e che all'evento positivo (accertamento di maggiori entrate) si accompagna l'evento di segno negativo degli effetti derivanti dalla predetta recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di detraibilità dell'IVA.

Signor Presidente, cari colleghi, sarò molto succinto. Questa mozione unitaria impegna il Governo a sostegno della candidatura della

ospitati, moltissimi a carattere istituzionale e religioso, hanno portato nella città migliaia di persone.

proprio come segno di una disponibilità e apertura da parte dell'arco delle forze parlamentari una verifica su un argomento come questo, su un impegno che interessa tutti e non soltanto uno schieramento, cioè su una sfida che riguarda Roma, una città che è di tutti e non soltanto di qualcuno

al comitato promotore ed organizzatore una direzione autorevole, rappresentativa dell'insieme del Paese

della struttura del comitato che dovrà seguire i passi successivi verso la candidatura sia sentito come un'organizzazione e un comitato promotore di tutti, che quindi, in qualche modo, sia in grado di rappresentare questo sforzo unitario. Mi auguro che, così come abbiamo

senatore Bettini, per l'illustrazione di questa mozione che rimette al centro il nostro Paese su questa straordinaria missione politica che dobbiamo compiere.

con la presentazione di questa mozione per la candidatura della città di Roma ad ospitare i trentunesimi Giochi olimpici e Paraolimpici del 2016, il nostro Paese tende ad ottenere che le Olimpiadi si svolgano in Italia ed è questo un momento importantissimo per il mondo sportivo, che trova l'impegno ed un preciso sostegno da parte di tutte le forze politiche. Si superano così, e non è cosa di poco conto, le diversità proprie della politica che, comunque, sono sempre frutto della democrazia. La presentazione delle due mozioni *bipartisan* alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è la migliore dimostrazione che maggioranza e opposizione sanno superare le loro differenze e collaborano nell'interesse reale del Paese.

quando si ha la certezza diffusa e condivisa della rilevanza dell'evento, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche dal punto di vista economico, sociale e turistico. Di ciò va dato atto a tutte le forze politiche che si riconosceranno in questo importante progetto. Il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive si occuperà di attivare ogni possibile iniziativa che consenta la candidatura di Roma come sede dei Giochi olimpici del 2016.

i Campionati mondiali di ciclismo a Mendrisio nel 2009, i Campionati mondiali di nuoto a Roma nel 2009, i Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2009, i Campionati mondiali di pallavolo a Roma nel 2010. Certamente le Olimpiadi estive del 2016 assumono un'eccezionale rilevanza e quindi è richiesta coesione, convincimento sincero. La mozione*bipartisan*

sia necessario operare con molta puntualità perché l'investimento sarà grande (circa 15 miliardi di euro) e perché dovremo superare la sfida di altre 17 città

tutto il Parlamento può però aiutare il successo di un lungo percorso che oggi è solo alla sua tappa iniziale.

è convinto della necessità di presentare una mozione così ampiamente sostenuta da moltissime forze politiche e anche da singoli senatori

Sapete che molti di noi sostennero la candidatura di Roma nel 2004,

Non vi fu quell'ampia convergenza perché il Paese non fu unito. Desidero sottolinearlo con molta chiarezza: vi erano, evidentemente, retropensieri, vi erano interessi per altre città.

dinamicità, che rimette in campo la nostra competitività, il nostro *appeal* come Paese a livello internazionale. Vorrei ricordare la straordinaria Olimpiade

si riescono a coinvolgere non solo le forze politiche e gli addetti ai lavori, ma anche le associazioni sportive, i gruppi di base dello sport e i gruppi dilettantistici, tanto più bisogna essere attenti

che non solo non creano problemi di impatto ambientale (che purtroppo, devo dire, si sono riscontrati anche per le Olimpiadi di Torino) ma che, invece, sono da questo punto di vista

la candidatura per mano: qualità progettuale, qualità nella partecipazione, qualità di un Paese che investe nella propria capitale. Se riusciremo a fare questo credo che questa volta otterremo un

Presidente, credo che, per l'ora intervenuta, sia il caso di cominciare a valutare la prosecuzione dei lavori anche per la settimana prossima. del decreto sugli sfratti non sia stato concluso. Pertanto, aver anticipato con il calendario corrente dei lavori la discussione dell'assestamento e del rendiconto a martedì mattina,

Lo faccio anche in base all'esperienza che ho potuto vivere come amministratore nel candidare la città di Torino e la Regione Piemonte alle Olimpiadi invernali del 2006. Anche in quel caso - e fu un fatto essenziale, anzi direi determinante - ci fu una consistente convergenza istituzionale sulla candidatura, come mi sembra e auspico avvenga pure in questa specifica occasione. Questo elemento

(estremamente importante, ma al contempo difficile perché i concorrenti sono veramente molto agguerriti) ci si debba presentare, nei confronti dei membri del CIO, con una convergenza istituzionale assolutamente compatta.

di acquisire la candidatura nei confronti di altre città che dal punto di vista della storia degli sport alpini molto più accreditate rispetto alla nostra. Il fatto che una città, un capoluogo, una capitale, si proponesse per lo svolgimento dei Giochi olimpici fu indubbiamente un elemento che fece pendere pendere a nostro favore la scelta dei membri del CIO. Credo che quelle di Torino - non è stato sufficientemente ricordato - siano state, nell'ambito delle Olimpiadi invernali, sicuramente delle Olimpiadi innovative. Infatti, una città, una capitale, un grande concentrato e una grande proposta culturale collegata all'evento sportivo hanno rappresentato sicuramente l'elemento di successo delle Olimpiadi di Torino. Chiaramente Roma non ha queste criticità perché di per sé è una città che offre, dal punto di vista culturale e turistico, una immensità di attrazioni. Bisogna mettere in evidenza nel *dossier* - credo che questo debba essere un monito anche relativo all'esperienza di Torino - la definizione degli impianti,

alla fine il risultato è che qualche impianto oggi non trova una sua utilizzazione e un suo equilibrio economico, tanto per intenderci: questi impianti rimangono sulle spalle delle

a chiedere una unità del Paese sulla candidatura di Roma. La candidatura di Roma mi ha fatto leggere, quando era ancora in corsa la città di Milano, di Milano, un grande egoismo da parte del sindaco Veltroni a volere ad ogni costo le Olimpiadi nella capitale.

da Monaco nel 1972: la Germania, la Repubblica federale tedesca, riconosce i princìpi di federalismo di cui noi siamo portatori ed esponenti, anche nella distribuzione sul suo territorio delle Olimpiadi.

Sappiamo che le Olimpiadi del 2012 sono assegnate alla città di Londra. Mai, nella storia moderna delle Olimpiadi,

Si vanno a comperare gli amici, i componenti del CIO del Terzo mondo, pagando le lauree ai loro figli, magari vicino alla Sorbona**,** e poi questi danno

Veltroni, e non solo Veltroni ma anche Petrucci, con l'invidia sul volto di volere ad ogni costo le Olimpiadi a Roma.

a Roma. E perché non farle a Bari? Basta con questo centralismo, noi non possiamo condividere questi princìpi prepotenti nei confronti del Paese Italia;

Dobbiamo fare anche una riflessione. Guardiamo agli atleti, quelli che portano a casa le medaglie; ma dove abitano questi signori? Vi siete mai chiesti da dove arrivano? Andiamo a vedere. Gli

per il bene di tutti cominciare ad affrontare la strada del federalismo. Mi rivolgo in particolar modo agli amici della sinistra: voi che siete riformisti, guardate che il centralismo è sempre più imperante. Lo vediamo anche

ad ospitare nel nostro Paese i Giochi olimpici - per sostenere la candidatura non solo italiana ma, soprattutto, della capitale d'Italia. Abbiamo sottoscritto questa mozione nella consapevolezza che tutti gli elementi che possono portare nel nostro Paese iniziative di carattere internazionale internazionale e, soprattutto, lo sport e i Giochi olimpici rappresentino un valore, un valore fondamentale per la convivenza civile tra i popoli. Credo che in questo momento storico l'Italia possa svolgere un ruolo importante (lo stiamo facendo e lo abbiamo fatto nel passato per la politica estera). In questo momento, candidare quasi all'unanimità il nostro Paese ai Giochi olimpici rappresenta un salto di maturità politica, che sottolinea il livello di una classe dirigente politica attrezzata;

una mozione che riscopre la vocazione italiana; è una mozione che candida Roma ad un ruolo importante. Questa volta, senatore Bettini - come lei ben sa - non muoveremo una critica al sindaco;

nella lettera firmata dal Presidente del Consiglio precedente, che dava questo *input*; ma, soprattutto, credo che la scommessa del Governo italiano - ed anche del CONI - di portare a casa, con il sostegno di tutte le forze politiche, un risultato così importante possa essere valutata, nei prossimi mesi, in termini favorevoli e positivi. Assicurare alla candidatura di Roma un supporto finanziario,

che sia funzionale non solo alla città di Roma, ma allo sport nella sua complessità. Che si ritorni, finalmente, anche grazie alla possibilità offerta da queste Olimpiadi, a valorizzare

in tutte le sedi, politiche e non, il supporto dell'UDC non solo a questa candidatura ma a tutti gli aspetti politici e organizzativi che possono dare, collega Bettini, quel valore aggiunto a un risultato che tutti noi auspichiamo.

Signor Presidente, noi voteremo a favore di questa mozione, che peraltro abbiamo sottoscritto.

dei volenterosi né di altri soggetti contro qualcuno, e sarebbe davvero risibile

una coalizione che allude a dialoghi o a confronti politici che non mi pare abbiano alcuna possibilità di essere confusi con la scelta, la scelta, seria e matura, di candidare la capitale del Paese a ospitare le Olimpiadi. di una determinazione a cui si è pervenuti attraverso varie fasi che sono state illustrate dal collega senatore e che io penso debbano essere considerate come tappe di avvicinamento ad un processo che mi auguro possa portare a un risultato positivo per Roma per Roma e per il Paese. Noi abbiamo una considerazione che vogliamo sottolineare e vorrei evitare che vi fossero delle strumentalizzazioni banali e politiche. Non sappiamo come saranno gli equilibri politici a Roma non si può proiettare sul 2016 la realtà politica di oggi, ma pensiamo invece che il ritorno a Roma delle Olimpiadi dopo 56 anni possa essere, e auspichiamo che sia, l'occasione anche per dare un segno possibile che le Olimpiadi, tornando nel vecchio continente, possano riabbeverarsi allo spirito delle fonti, quindi a qualcosa che abbia molto a che fare con lo sport, il confronto, la solidarietà, la partecipazione, la crescita culturale, lo scambio, e molto meno con quanto di gigantismo economico si è determinato nel corso degli ultimi anni. Se osserviamo che cosa sta succedendo a Pechino

ci si interroga e si viene interrogati sulle conseguenze sul piano sociale, dell'equilibrio della città e del rapporto e del rispetto del territorio. Da questo punto di vista penso che noi, nel sostenere la candidatura, come dobbiamo, con la coralità con cui abbiamo firmato la mozione che adesso andiamo a votare,

virtuoso da questo punto di vista, ma c'è ancora molto da fare. Dobbiamo considerare il traguardo delle Olimpiadi come occasione di ricucitura del centro e delle periferie,

Dobbiamo considerare il traguardo delle Olimpiadi come occasione di una crescita

permanentemente presente il rapporto tra lo sport e la società. Non è dato pensare ad una crescita di risultati sportivi e anche di elementi di eccellenza nello sport in una società che non cresca dal punto di vista della qualità della vita. Dobbiamo determinare una condizione in cui la crescita e lo sviluppo dello sport corrispondano ad una crescita della qualità della vita a Roma, nell'*hinterland*, nell'area metropolitana e nella Regione,

Dovremo stare molto attenti affinché gli *sponsor* non prendano la mano allo sport.

e quindi anche il rapporto tra società e potere. Credo che le Olimpiadi a Roma possono costituire, da questo punto di vista, un'occasione ed un terreno utile affinché, a partire dalla cultura di questo Paese (mi auguro con la partecipazione culturale di tutte le forze che in Italia si sono sviluppate),

Signor Presidente, siamo così pochi che ci possiamo permettere qualche digressione, per questo mi perdoni se la prenderò un po' da lontano. Appena è emersa la candidatura di Roma per ospitare le prossime le prossime Olimpiadi si è fatto vivo il solito scetticismo all'italiana e ci si è chiesto: sarà Roma nella condizione di organizzare un evento che si è fatto così complesso, che richiede strutture e tutta una serie di attenzioni e di mezzi? Il nostro Paese, che tra l'altro non attraversa un periodo particolarmente felice dal punto di vista delle risorse economiche e finanziarie, sarà in grado mai di sostenere un'impresa di questa natura? natura? A parte il fatto che non ho mai visto un pessimista giovare a qualcuno o a qualcosa, ritengo che abbiamo molti motivi per credere in ciò che facciamo quando sosteniamo questa candidatura. Consentitemi

persino quella parte, che oserei definire laica nella sua irritualità, dell'elogio del Papa. Fu un consenso così straordinario, diffuso e condiviso che ci parve di poter credere che eravamo un Paese in grado di far fronte ad un impegno di quella natura. Rispetto ad allora le condizioni di oggi sono cento volte più idonee. Presidente, la guardavo prima mentre un suo corregionale parlava delle Olimpiadi e mi pareva di poterle essere almeno questa volta complice nel credere che lei stesso potesse dissentire dall'idea che Roma stia compiendo un'operazione truffaldina, qualcosa di di intollerabile e inconfessabile ai danni del Paese. Siamo in un momento in cui possiamo compiacerci di aver trovato in quest'Aula, ad esempio, una straordinaria unanimità nel mettere insieme le idee che ci devono condurre a questo traguardo con animo condiviso, in cui ciascuno può mettere del suo affinché questa cosa riesca nel modo migliore possibile. D'altronde, Torino ha dato già questa prova.

sono felice se in quest'Aula finiranno per prevalere le idee delle persone di buona volontà, che non vivono di *slogan*, che non sono animate da pregiudizi,

Signor Presidente, colleghi senatori, anch'io sono tra i firmatari della mozione e il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di essa. D'altro canto, l'iniziativa è partita proprio dall'amico e collega Alemanno alla Camera. Tuttavia, credo che qualche considerazione politica vada spesa per porre un limite e per perimetrare il senso di questa convergenza; credo altresì che, prima di fare qualche considerazione politica, se non altro per amore di verità

Roma, come ha sottolineato il collega Bettini, rimane oggettivamente l'unico candidato in campo che abbia le infrastrutture, invero un po' antiche, collega Bettini, perché risalgono al 1960 e al 1990

Vorrei aggiungere una considerazione sul perimetro della convergenza, per amore di verità. Lo dico con il massimo rispetto e la massima simpatia per chi mi ha proceduto: voglio solo ricordare che la Germania federale, nel 1972, fece le Olimpiadi a Monaco e non a Berlino sì per un senso di federalismo, ma anche e soprattutto perché Berlino non era più la sua capitale, che in quel momento era Bonn. Quindi, la Germania federale avrebbe avuto qualche difficoltà

per mettere davvero le ali a questa candidatura. Bene, la mozione è chiara: ci occorrono l'attenzione e le risorse del Governo, ma ci occorre anche qualcos'altro,

e nelle mobilitazioni di appetiti e di attenzioni che ci furono intorno a quegli avvenimenti. Credo che questo sia il primo passo: una grande discussione su come vorremmo interpretare tale scadenza. Il secondo punto è quello di superare quella che possiamo definire

Temistocle aveva l'abitudine di chiedere l'aiuto degli oppositori e di Aristide soltanto quando stavano arrivando i persiani con le loro navi; per tutto il resto della normale vita politica di Atene li teneva in esilio.

di affrontare i grandi problemi e i grandi ritardi che ci sono, mettendoli al centro del dibattito e non negandoli e nascondendoli dietro boa di struzzo e scintillanti quanto effimeri avvenimenti culturali, che pure hanno la loro importanza. Tale salto di qualità è importante e necessario, preliminarmente necessario, e in questo ci può essere un'autenticità di rapporto tra maggioranza e opposizione. Aggiungo che è necessario un altro grande sforzo collettivo.

sulla discussione di questa mattina e sul conseguente voto, che mi auguro possa veramente coinvolgere

accomunare tutti anche la volontà di giungere alla meta nell'interesse non soltanto dello sport italiano perché quando parliamo di sport italiano parliamo dell'intera

pensare. Se è vero che quest'Assemblea votò tutti gli emendamenti e tutti i provvedimenti di carattere legislativo per sostenere opportunamente, a candidatura andata a segno, quindi ad Olimpiadi ottenute nel caso di Torino - e il collega Ghigo ne ha già fatto riferimento - credo che ora tutta l'Assemblea partecipi a considerare il provvedimento in discussione

2020. Inoltre, Pescara è sede dei Giochi del Mediterraneo del 2009, la città lo volle e spero che risolva problemi di carattere politico locale che ancora non fanno decollare l'organizzazione. Sarebbe il caso che il Governo vi riponga, come mi risulta stia facendo, tutte le dovute attenzioni. Altre città saranno sede di importanti avvenimenti, così come altre lo sono state in questi anni.

Torino, per le Olimpiadi estive e invernali precedenti, lo sarà nell'eventualità che Roma possa ospitare le Olimpiadi nel 2016.

attestandosi al 4 per cento; successivamente, è ancora cresciuto fino al 2004-2005, attestandosi al 4,5

vive problemi tipici di tutta l'Europa, ma che ha elementi di sviluppo sorprendenti se li paragoniamo alla situazione di dieci anni fa. quindi che un voto favorevole che unisca tutto il Parlamento sia un atto dovuto.

Presidente, signor rappresentante del Governo, signori colleghi, la candidatura della città di Roma come sede dei Giochi olimpici del 2016 è una candidatura condivisa, sostenibile, utile e competitiva. È per questa ragione che la mozione in votazione, sulla quale abbiamo visto convergere numerose adesioni trasversali della maggioranza e dell'opposizione, rappresenta per tutto il Parlamento italiano un motivo di particolare soddisfazione. Ci piace credere che questo metodo possa essere adottato, signor Presidente, anche per altre grandi battaglie che riguardano il nostro Paese e la città di Roma, la capitale d'Italia, a cominciare dalla finanziaria e dai fondi per Roma Capitale. La richiesta rivolta al Governo di garantire il sostegno, soprattutto economico, alla candidatura di Roma ad ospitare i Giochi olimpici sappiamo che è molto impegnativa, visto che ci muoviamo entro margini di finanza pubblica purtroppo ristretti, a fronte di un'entità ragguardevole di cifre da mobilitare. Sappiamo anche che i passaggi per arrivare alla scelta finale del Comitato olimpico internazionale (CIO) sono ancora lunghissimi: il prossimo luglio il CIO invierà il *dossier* sulla candidatura; a gennaio 2008 il CONI ufficializzerà definitivamente la scelta di Roma; a marzo 2008 il CIO sceglierà, tra le 18 richiedenti, le cinque città che parteciperanno alla corsa finale; nel dicembre 2008 i candidati dovranno inviare al CIO il *dossier* definitivo e, infine, a Copenaghen, nel settembre del 2009 il CIO sceglierà la sede dei Giochi del 2016. Senatore Leoni, settembre del 2009 è dunque il momento in cui avverrà tale scelta. Voglio dire ai colleghi della Lega Nord che tale data non è compatibile con le accuse di strumentalità della decisione, finalizzata a campagne elettorali che non ci sono in quel periodo. le elezioni europee si saranno già svolte da tre mesi, le elezioni regionali arriveranno nove mesi dopo, le elezioni politiche un anno e otto mesi dopo. Lei insulta l'intelligenza degli italiani se pensa che la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2016 sia utilizzata a fini elettorali. Riuscire a portare i Giochi olimpici a Roma crediamo sia per tutti un grande sogno: un'ambizione a cui la maggioranza e l'opposizione, responsabili, vogliono puntare con tutte le loro forze; un'ambizione impegnativa, ma non impossibile. A fronte dei 17 rivali da contrastare, Roma ha ottime carte da giocare: 22 impianti già pronti, 20.000 unità ricettive già in opera, senza contare le strutture che resteranno in eredità dei Giochi olimpici dai mondiali di nuoto e di pallamano, nonché di pallavolo, che si terranno, rispettivamente, nel 2009 e nel 2010. Roma non parte da zero e già negli anni scorsi ha dimostrato di essere capace di ospitare grandi eventi sia civili, sia religiosi. Penso, signor Presidente e signor Sottosegretario, ad esempio, ai giorni che hanno preceduto e accompagnato le solenni esequie di Giovanni Paolo II, quando circa tre milioni di pellegrini stranieri e di connazionali sono giunti nella capitale. In quell'occasione accadde qualcosa di particolare, di straordinario: come se un'altra Roma avesse improvvisamente preso vita dentro Roma stessa. L'esempio di civiltà e ordine e ospitalità che questa città ha dato al mondo intero è ancora impresso nei nostri occhi. Le forze politiche che hanno presentato la mozione che ci apprestiamo a votare testimoniano che questa candidatura è un atto di civiltà, un atto di grande forza per Roma, indipendentemente dalle ideologie e dalle appartenenze politiche, senatore Leoni. Siamo tutti consapevoli che questa candidatura rappresenta il recupero di centralità della città, rispetto a tutte le dinamiche nazionali. Lo hanno affermato, oltre al collega Bettini, il senatore Baccini, il senatore Augello, solo per citare alcuni fra i tanti colleghi favorevoli a questa mozione. Voglio anche dire che tutto il Parlamento italiano, sia la Camera sia il Senato, salvo alcune eccezioni, ha appoggiato questa candidatura, come ha appoggiato quella di Torino, dove si sono svolte eccellenti Olimpiadi invernali, indipendentemente dai soggetti che le hanno approvate a suo tempo. Ciò detto, a quanti hanno, più o meno, esplicitamente palesato riserve o malumori rispondiamo che tanto più si esaltano le autonomie, tanto più un federalismo virtuoso deve avere nella propria capitale un simbolo dell'unità della Nazione. E questo ne è un bell'esempio. Per il buon esito finale va tuttavia rilevato che non basterà l'impegno del Governo, ma sarà fondamentale, nella presentazione del *dossier* per Roma, la presenza di forti e durevoli garanzie finanziarie per coprire gli investimenti, visto che la massima manifestazione sportiva richiede conferme continue, oltre che ingenti. Per ospitare i Giochi olimpici, la capitale dovrà affrontare una competizione difficile, che le istituzioni possono e vogliono sostenere per riuscire a tagliare questo prestigioso traguardo.

auspicando che essa trovi in quest'Aula la più larga approvazione possibile. La candidatura di Roma a sede delle Olimpiadi 2016 rappresenta di per sé il primo, importante gradino

signor Presidente. aderisco alle motivazioni di contrarietà esposte dal senatore Leoni, ma ritengo vada aggiunto dall'altro. Con un linguaggio lieve, quasi suadente, si vuol far credere che quella delle Olimpiadi a Roma sia una questione di pura sportività, di pura solidarietà, sotto il profilo dell'appartenenza della Capitale al sistema Italia. Noi, viceversa, vediamo in questa operazione la ripetizione dell'operazione 1960,

del secolo scorso, che fece emergere una nuova categoria economica, un nuovo ceto imprenditoriale, che condizionò poi la politica di Roma e del Paese intero. Un ceto imprenditoriale che uscì dal nulla attraverso la realizzazione di Roma EUR. Passarono i Giochi olimpici e rimase quel ceto imprenditoriale; rimasero e rimangono, tuttora, gli effetti dell'improvvida insorgenza di quella nuova classe economico-imprenditoriale.

sentivo girare ieri sera la voce di una richiesta di votazione elettronica. I colleghi della Lega hanno espresso con coerenza le loro ragioni, che non condivido. non condivido. Chiedo loro di evitare che questa mozione si debba votare martedì prossimo, perché comunque si voterebbe.

richiedere, insieme a 12 colleghi, la verifica del numero legale. Stiamo parlando di Olimpiadi che si svolgeranno non a Roma - se vi si svolgeranno - ma in Italia.

tale importanza. Voi portate a casa il risultato di aver dimostrato che l'Aula è vuota mentre si vota questa mozione; consentiteci però di farla passare. Questa procedura usiamola nel momento della coerenza, quando chiederemo al Governo

Colleghi, la mia esperienza mi dice che neanche votare per quattro porterebbe a risultati diversi. Dichiaro chiusa la votazione.

come è già stato annunciato - tra i Capigruppo, la seduta antimeridiana di martedì 24 ottobre non avrà luogo, per consentire alle Commissioni competenti di proseguire nell'esame dei provvedimenti previsti dal calendario, con particolare riguardo al decreto‑legge in materia di emergenza abitativa.